L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge

Presidente, apprendiamo con sorpresa la decisione del relatore, perché questo provvedimento, che può apparire di poca importanza per i colleghi senatori residenti in Italia, è di grande importanza per la comunità italiana all'estero, come ho ricordato questa mattina.

oggi abbiamo lavorato per cercare questi punti d'incontro non semplici, perché anche nella mia parte politica vi sono opinioni divergenti su alcuni punti di questo disegno di legge. Abbiamo, però, davvero compiuto un grande sforzo

dove siano i problemi. Come opposizione, noi abbiamo affrontato le nostre difficoltà ed eravamo pronti a votare gli emendamenti. Mi preme poi ricordare un punto importante, soprattutto all'indirizzo del Governo.

Patria. Volevo ricordare al Governo che questa mattina ho precisato che, come Gruppo del Partito Democratico,

Noi chiediamo formalmente un impegno del Governo affinché, come già è stato comunicato al Consiglio generale degli italiani all'estero, in primavera, e non alla fine dell'anno, si vada al

Ribadisco in quest'Aula, a nome del Governo, che entro il 31 dicembre 2012, come prevede la legge, procederemo all'elezione dei COMITES. Se questa legge nuova di riforma, alla quale tutti i Gruppi parlamentari hanno intensamente lavorato, sarà pronta, questo avverrà secondo le regole che verranno stabilite con la nuova legge, altrimenti con la legge esistente procederemo all'elezione dei COMITES nel 2012.

breve e di buon senso. Ritengo, quindi, doveroso, anche per il tipo di lavoro che si è svolto in questi lunghi mesi, non far partorire gattini ciechi per la fretta, e quindi accogliere la proposta del relatore.

***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007***

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta

Signor Presidente, il provvedimento in esame riproduce il testo dell'analogo disegno di legge presentato nella scorsa legislatura (Atto Senato n. 884), su cui la Commissione esteri, previo parere favorevole delle Commissioni e parere non ostativo della 5a Commissione, si era espressa favorevolmente già l'11 ottobre 2006, venendo successivamente approvato dall'Assemblea il 13 febbraio 2007. Ricordo tuttavia che, nell'ambito dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento, l'esame della Commissione affari esteri e comunitari dell'Atto Camera n. 2265 non è giunto a conclusione. Il provvedimento in esame assume un significativo rilievo sotto il profilo economico-culturale e politico. Il rilievo economico-culturale è dato dalle prospettive di apertura del mercato cinese alla produzione cinematografica italiana, nonché dalle potenzialità che tale *partnership* è in grado di offrire alla produzione italiana, tenuto conto - da un lato - della vivacità della produzione cinematografica cinese, che nel recente passato ha conseguito anche significativi riconoscimenti nelle manifestazioni culturali internazionali, e - dall'altro del fatto che in passato diverse produzioni italiane sono state realizzate in Cina e la definizione dell'Accordo potrebbe consentire in futuro di disporre di maggiore sostegno *in loco*, ivi compresi possibili contributi cinesi. Sotto il profilo politico, tenuto conto che alla ricca produzione ufficiale si accompagna una significativa produzione cinematografica da parte di operatori cinesi, i quali tuttavia non possono produrre e diffondere le loro opere *in loco*, ovvero sono soggetti a pesanti restrizioni, è auspicabile auspicabile e probabile che un'intensificazione della cooperazione culturale in questo campo con l'Italia porti, come risultato ineluttabile, ad una maggiore apertura di quel Paese in termini di rispetto dei diritti civili e politici. Il disegno di legge reca la ratifica di un Accordo che si propone di realizzare un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca ed essere competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi. Nel merito, l'Accordo precisa il significato di "film in coproduzione" e stabilisce che ogni film coprodotto goda degli stessi vantaggi dei film nazionali. Vengono poi individuati i requisiti che i coproduttori devono possedere, fissando alla quota del 20 per cento del costo totale del film l'apporto minimo al progetto di coproduzione. Si stabilisce che il personale, artistico e tecnico, impiegato nella coproduzione debba essere di cittadinanza italiana (inclusi i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea) o cinese (inclusi i cittadini di Hong Kong e delle Regioni ad amministrazione speciale di Macao), e che tale personale è tenuto a rispettare la legislazione vigente, gli usi, i costumi e il credo religioso del Paese in cui le riprese hanno luogo. Ulteriori norme autorizzano inoltre 1'ingresso di cittadini dell'altro Paese e la temporanea importazione di attrezzatura cinematografica nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché lo svolgimento di riprese in Paesi terzi laddove la sceneggiatura o l'azione dei film lo rendano necessario. alla negoziazione fra i coproduttori sono quindi rimesse sia le decisioni riguardo all'accesso dei film in coproduzione ai festival internazionali sia la ripartizione dei proventi derivanti dai diritti d'autore, i quali appartengono ad entrambe le parti contraenti. L'Accordo dispone che i film coprodotti debbano essere esaminati ed approvati dalle autorità competenti dei due Paesi individuati dall'Accordo stesso, precisando che gli stessi possono essere distribuiti e proiettati in pubblico, all'interno e all'esterno di ciascun Paese, solo dopo il rilascio del relativo permesso da parte delle rispettive autorità competenti. Tale ultima disposizione, contenuta all'articolo 10, è stata oggetto di un approfondito dibattito nel corso dell'esame del Trattato da parte della Commissione esteri della Camera dei deputati nel corso della scorsa legislatura e anche da parte della Commissione esteri del Senato.

dell'articolo 10, volta ad evitare eventuali interventi autorizzatori da parte delle Autorità cinesi, che avrebbero potuto delineare una forma di censura incompatibile con l'ordinamento italiano. Tale nota infatti prevede che l'approvazione provvisoria data a sceneggiatura e progetto filmico non possa essere ritirata ad opera conclusa, salvo che l'opera completata si discosti in maniera sostanziale dal progetto approvato. È stato altresì stabilito un meccanismo di automatismo tra approvazione definitiva e concessione del permesso di uscita nelle sale; di uscita nelle sale. La Commissione, nel corso dell'esame, ha altresì analizzato una proposta di ordine del giorno relativo ad un impegno del Governo a monitorare con attenzione, nell'attuazione dell'Accordo, eventuali operazioni di censura sulle opere cinematografiche. In conclusione, la Commissione propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Perché? Perché, nonostante si tratti di un Accordo importante - in generale, sono importanti gli accordi che stabiliscono relazioni e cooperazioni culturali tra i Paesi,

di cooperazione culturale con un altro grande Paese produttore come l'India, e nulla di questo apparato censorio compariva in quell'Accordo. Per questo si apriva un problema di principio, che riguardava sia la compatibilità di quell'intesa con il nostro quadro costituzionale di libertà, che veniva coinvolto in strutture di censura incompatibili con il nostro ordinamento e, prima ancora, con la nostra cultura,

Come il relatore ha ricordato, il Governo, sulla base di quella discussione e di quella richiesta di riesame, ha proceduto a negoziare con le autorità cinesi una nota interpretativa dell'articolo 10 del Trattato, che discute ed interviene sugli aspetti censori.

possibilità di equivoci interpretativi, con tutto ciò che ne consegue. Per questa ragione, in occasione della discussione odierna e per trovare uno sbocco a una situazione che andava in qualche misura risolta e di un accordo che andava

Paese e nel nostro Parlamento ma più in generale, una riflessione su quale rapporto debba esserci fra interessi e principi, fra accordi ispirati a un concreto realismo ed elementi che riguardano la difesa di un quadro di principi che non può essere fatto valere solo nelle occasioni più drammatiche come quelle che oggi si stanno verificando, ad esempio, nel quadro mediterraneo. Per questo motivo,

una discussione che non nasconda i problemi, che non pensi che le relazioni diplomatiche debbano essere subordinate al tacitamento delle questioni che separano e dividono le differenti visuali e valutazioni dei problemi,

Signor Presidente, chiedo scusa per questo leggero ritardo, ma tanto questo Trattato quanto il prossimo relativo al Libano sono stati licenziati pochi minuti fa dalla 3a Commissione, non consentendo la presentazione di documenti a corredo del nostro dibattito. Ho ascoltato l'illustrazione dell'ordine del giorno G100 da parte del senatore Marcenaro e gli chiedo se posso aggiungere la mia firma,

la quale non soltanto ha disertato la cerimonia per la consegna del premio Nobel, argomento che ci ha interessato (come ricordava poco fa il senatore Marcenaro, i maggiori Gruppi parlamentari hanno presentato delle mozioni per un dibattito urgente), ma addirittura ha escluso Liu Xiaobo dal contatto con i familiari e con il resto del mondo. Che tipo di censura

credo Falun Gong, per non parlare di tutta una serie di interpretazioni del confucianesimo, che non necessariamente siamo tenuti a conoscere.

unico? Si può non porre la questione dell'imposizione dell'aborto di Stato da parte di Pechino, ormai da trent'anni a questa parte, come possibile oggetto di una coproduzione televisiva? Io credo che siano tutte questioni che si devono porre all'attenzione di un rapporto franco e sano con un Paese, che è sicuramente importante, ma che altrettanto sicuramente non garantisce un diritto umano che sia uno, anche se si tratta di cinesi:

i film in coproduzione devono essere approvati dalle competenti autorità dei due Governi. L'autorità competente per il Governo della Repubblica italiana è il Ministero dei beni culturali, mentre l'autorità competente per il Governo della Repubblica cinese è una

Un Paese che ha bloccato l'accesso alla posta di Google, che ha bloccato Facebook, che continua a bloccare Internet ogni volta che c'è la necessità di non far sapere che alcune cose vanno male, dubito che conferisca al Ministero per le attività culturali il potere di coprodurre potere di coprodurre dei film che hanno a che fare con argomenti particolarmente sensibili. «I produttori e gli studi cinematografici coinvolti», recita l'articolo 3, «nelle coproduzioni tra i due Paesi devono avere personalità giuridica». Quindi, ancora una volta, devono passare molto probabilmente dal Ministero dell'interno della Repubblica popolare cinese. All'articolo 5, si dice che «La proporzione del *cast* tecnico e artistico di ciascuna parte dovrà essere negoziata tra i due produttori, nel rispetto della sceneggiatura, prima che il progetto venga sottoposto all'approvazione delle competenti autorità di entrambe le parti. Anche senza gli apporti tecnici e artistici, le coproduzioni solo finanziarie sono consentite». Ancora una volta, il valore artistico è messo da parte: occorre mantenere le quote. che «Le riprese in esterni in un Paese che non partecipa alla coproduzione possono essere autorizzate se la sceneggiatura o l'azione del film lo renda necessario e se i tecnici di una o di entrambe le parti partecipano alle riprese». L'articolo 8 dice che «Il personale di entrambe le parti impiegato nella coproduzione dovrà rispettare la Costituzione, le leggi e i regolamenti, le culture etniche, il credo religioso e gli usi e costumi locali del Paese in cui hanno luogo le riprese in esterno». Posto che si faccia in Italia, i problemi della non applicazione, anzi, della violazione quotidiana della Costituzione italiana i Radicali li ripetono tutti i giorni, ma se si dovesse andare a fare in Cina, dove in effetti uno dei primi articoli della Costituzione riconosce i gruppi etnici e affida loro dei diritti particolari di autogoverno e si dovesse tenere a mente, però, cosa questo Parlamento molto spesso con delle risoluzioni ha adottato relativamente alla situazione in Tibet, credo che ancora una volta la risposta corale che dovrebbe scaturire è un no a questo tipo di contratti, perché chiaramente sappiamo che i milioni di tibetani in Tibet, le decine di milioni di uiguri nel Turkestan orientale o in cinese Xinjiang, per non parlare dei pochi manciuri e mongoli rimasti, sicuramente non godono di una che sia una autonomia in virtù del loro non essere etnicamente han. L'articolo 10 è stato più volte ricordato: una volta ultimato un film cofinanziato - quindi, attenzione, una volta ultimato - e prodotto congiuntamente, deve essere un'altra volta esaminato e approvato dalle competenti autorità,

seminato. In ultimo, l'articolo 14 riprende i dubbi relativamente a chi per i cinesi dovrebbe prendere in considerazione l'applicazione di questo Accordo.

esamineranno» (ancora una volta) «l'applicazione del presente Accordo e si adopereranno per risolvere ogni problema che insorga nell'applicazione stessa». Gli altri articoli sono stati ricordati, giustamente, ottimamente, dall'ordine del giorno G100 presentato dal senatore Marcenaro.

predica del rispetto dei diritti umani - ripeto: diritto alla vita, diritto alla libertà religiosa, diritto alla necessità di tenere di conto delle esigenze di gruppi etnici, primi fra tutti i tibetani, a favore dei quali il 10 marzo questo Parlamento da anni, avendo anche il più grosso gruppo interparlamentare di sostegno al popolo guidato dal Dalai Lama, si richiama

Accordo, qualora venisse oggi ratificato, non diventeranno mai operative, perché non sarà possibile fare altro che quotidianamente discutere tutta una serie di scelte, a meno che non si voglia fare una serie monografica su quanto è alta la Torre di Pisa o su quanto pende, su quanto sia larga la Piazza Rossa, o eventualmente partecipare - come già, ahinoi, avviene in Patria - alla riscrittura del divino Celeste è un preoccupantissimo precedente che i colleghi senatori, se hanno prestato attenzione a questo piccolo intervento, si mettono sulla coscienza. Ci sono 1.300 milioni di persone che non godono di una libertà che sia una. Dare la libertà al Governo di poter ancora una volta silenziare una minima voce che possa sollevare il dubbio che la Costituzione cinese vada bene com'è credo sia una responsabilità molto grave che viene assunta oggi.

anticipato, quanto all'ordine del giorno presentato dal senatore Marcenaro, per quanto mi riguarda,

in Commissione per arrivare anche a tale impegno. Quindi, si è d'accordo sia per quanto riguarda la *ratio* che porta alla presentazione di questo ordine del giorno sia evidentemente per quanto riguarda il suo contenuto. il suo contenuto. Ovviamente, condivido anche molte altre osservazioni che il collega ha espresso in sede di discussione generale, non ultima tutta la cronistoria, corretta, precisa e puntuale di questo provvedimento. Per quanto riguarda quanto sottolineato dal senatore Perduca, non si può evidentemente che concordare sul fatto che la Cina presenta delle problematicità per quanto riguarda la violazione dei diritti umani. Esistono però due tipi di atteggiamenti: quello della chiusura e quello del dialogo. Ecco, ritengo che questo provvedimento, unito all'ordine del giorno del senatore Marcenaro, rappresenti proprio questa seconda proprio questa seconda strada, e che quindi anche di fronte a delle problematicità con la «P» maiuscola si possano ottenere maggiori risultati percorrendo la via del dialogo.

anche se questo rende perplessi forse è una ragione in più per cercare di percorrere tutte le vie che ci portano a rafforzare i rapporti e i mezzi

anni che i Radicali assieme al Dalai Lama chiedono a Pechino l'apertura di un dialogo per una soluzione politica che garantisca l'autonomia (e non l'indipendenza) di quella Regione, preservando tradizioni, culture e anche orientamenti religiosi millenari.

seguire alcuni provvedimenti, quando non si è necessariamente d'accordo. In questo caso, la vigilanza sarà radicale affinché l'ordine del giorno G100 venga rispettato, perché siamo nettamente contrari a questo provvedimento.

Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra l'Italia e il Qatar sottoscritto il 14 gennaio 2007. Esso risponde principalmente alle esigenze di provvedere alla mancanza di un Accordo di cooperazione culturale fra i due Paesi; stimolare iniziative nel campo della collaborazione culturale, ad ogni livello; adattare i contenuti dell'Accordo ai nuovi bisogni culturali, scientifici e tecnologici, nonché alla crescente importanza che essi stanno assumendo nelle relazioni internazionali. Tra gli aspetti qualificanti dell'Accordo giova richiamare la previsione di un proficuo scambio di informazioni culturali ed iniziative attraverso biblioteche nazionali ed istituzioni culturali

Sono previsti altresì scambi di inviti in occasione dell'organizzazione di festival ed altre manifestazioni culturali (articolo 3);

l'istituzione di una commissione mista per la realizzazione dell'Accordo e la promozione e lo sviluppo della collaborazione culturale (articolo 5). L'approvazione dell'Accordo avverrà conformemente alle procedure costituzionali in vigore presso ciascun Paese ed esso entrerà in vigore alla ricezione della seconda notifica

Vorrei ricordare la missione compiuta da una delegazione della Commissione affari esteri in Qatar nel gennaio 2010, alla quale ho partecipato anch'io, che ha permesso di approfondire la situazione politica, economica e sociale del Paese. In conclusione, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Vorrei ricordare che stiamo parlando di un Accordo di cooperazione culturale con il Qatar, ossia l'emirato nel quale ha sede Al Jazeera, il più importante strumento di comunicazione di massa del mondo arabo, che sta avendo in questo momento un ruolo assolutamente da protagonista in quello che

***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e

più tranquillo di quanto non lo siano stati quelli precedenti. Si tratta di uno degli accordi standard per evitare la doppia imposizione e segue quei noti schemi proposti dall'OCSE: è un provvedimento di 31 articoli, molto tecnico. Ricordo solo che la Convenzione tra Italia e Libano è stata approvata nel 2000, quindi sono passati più di dieci anni

solo che si segue lo schema consueto di far pagare le imposte alle persone nel luogo di residenza

solo per ricordare che questo trattato è stato firmato nel 2000 e che il Libano del 2011 è probabilmente diverso da quello del 2000, anche perché ha visto non soltanto un conflitto armato, ma anche la nostra presenza militare.

e non tutti possono essere sempre presenti nelle Commissioni dove vengono affrontate le questioni; fortunatamente, il senatore Marcenaro ha preparato un documento fondamentale per il trattato

Oggi la Siria, per l'appunto, va contro tutto ciò che era stato posto all'attenzione del Governo in quell'ordine del giorno, in cui gli si chiedeva di assumere tutta una serie di iniziative che, se dovessi

Desidero solo dire che ha ragione il collega Perduca: le ratifiche procedono con eccessiva lentezza, come abbiamo già denunciato altre volte. Questo è un problema innanzitutto del Governo: non di questo Governo ma, in generale, dell'istituzione Governo, che procede al concerto tra i Ministeri con troppa lentezza. Da ultimo, la scelta del Partito Democratico di chiedere il voto elettronico è stata una scelta, ovviamente, non di natura ostruzionistica, ma per riaffermare la dignità parlamentare delle ratifiche.

confermare il voto favorevole del Gruppo del PdL su questo provvedimento e anche per ricordare che, se è vero che procediamo con lentezza, magari anche troppa, alla ratifica di questi provvedimenti, ogni ratifica

domani è l'ultimo giorno di lavoro per 1.240 lavoratori dell'INPS che hanno un rapporto di lavoro di somministrazione e svolgono pratiche importanti e decisive per le attività dell'istituto. Questo in virtù del fatto che la manovra di luglio ha tagliato, come è noto - in modo selvaggio e senza discernimento la spesa pubblica. Ora, questi 1.240 lavoratori domani smetteranno di lavorare. Ho chiesto al Ministro che cosa intende fare e non ho ricevuto risposta. Alla Camera oggi sembra abbiano votato in Commissione lavoro all'unanimità una mozione che dovrebbe impegnare il Governo a risolvere il problema. Rimane il fatto che al Senato non si risponde - e su questo potrei sorvolare

riguarda oltre 1.200 lavoratori. La Presidenza si attiverà perché vi sia una risposta da parte del Governo. In ogni caso, penso che il tema possa essere

sui temi delle donne e della pace in riferimento alle azioni previste dalle Nazioni Unite, che aveva le firme necessarie per essere trattata con urgenza, come previsto dal Regolamento.

Signor Presidente, ritorno su molteplici interrogazioni ed interpellanze che ho presentato al Ministero dell'economia riguardanti la crisi sistemica, la speculazione dei banchieri con i prodotti derivati, pari ad oltre 600.000 miliardi di dollari, quelli negoziati fuori dai mercati regolamentati, cosiddetti *over the counter*. Oggi leggiamo che la crisi del credito

di fronte al Parlamento, di fronte al Senato e ai senatori, a fronte di circa 30 tra interrogazioni e interpellanze parlamentari, non dare uno straccio di risposta.

a fare i banchieri, così come Assogestioni - la società del risparmio gestito - che froda i risparmiatori, perché non si ottiene nulla da coloro a cui si affidano i fondi comuni di investimento.